Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

che negli anni sono degenerati fino a diventare veri e propri carrozzoni nei quali inserire un po' tutto. Avevamo anche convenuto sulla necessità di una riflessione

c'è altro esempio nella vita parlamentare italiana. Infatti, in questa materia, come in altre, la quantità fa anche la qualità e la quantità di questo tipo di maxiemendamento ha travolto travolto e stravolto qualsiasi regola e qualsiasi principio in materia di procedure parlamentari. L'invito che era stato rivolto alla Presidenza, quindi, era quello di avviare un dibattito negli organi competenti o, al limite, con una

non si sa come (ne discuteremo naturalmente in corso di seduta), vi è una valanga di provvedimenti - almeno si annunciano tali - che potrebbe costituire ulteriore occasione per ripetere quella procedura.

per altre questioni introdotte nell'agenda politica o già giacenti in Senato o nell'altro ramo del Parlamento. Mi riferisco, per esempio, alla tematica servizi pubblici locali, che tra l'altro è oggetto di un disegno di legge delega che addirittura - come è stato affermato anche da autorevoli esponenti del centro-sinistra con incarichi istituzionali - potrebbe confluire in questo decreto-legge o in qualche treno

quel dialogo che si è cercato di aprire tra maggioranza e opposizione su tanti temi (non ultimi la legge elettorale e la riforma costituzionale) sia i rapporti di

processo abrogativo di una norma. Quando le fonti normative non sono uguali ed omogenee, come si dice con termine giuridico, non c'è problema, perché una fonte superiore sovrasta una fonte inferiore, la legge è legittima perché c'è una norma costituzionale che la rende tale. Qui noi ci troviamo di fronte a due fonti normative omogenee: l'emendamento di cui si parla nella legge finanziaria e il decreto‑legge. e il decreto‑legge. Sul contenuto siamo d'accordo, va soppresso, ma abbiamo il timore che la procedura che si sta seguendo nell'approccio a questa norma non sia sufficiente a risolvere il problema. Vede, signor Presidente, quando le fonti normative sono omogenee, dello stesso grado, non vale più il principio gerarchico ma quello cosiddetto cronologico: una norma non può abolire una volontà di fare una cosa diversa,

il Presidente della Commissione bilancio della Camera per rispondere a quell'esigenza che fu largamente sottolineata. Naturalmente il lavoro, prima in Commissione e, se servirà, anche in Aula, si svilupperà con il rilievo che deve avere un impegno di tal genere, assunto con tale solennità dalla nostra Aula e poi ripreso anche dal Capo dello Stato. Quindi, vi assicuro che la cosa non è ferma, sta andando avanti ed avremo occasione di discuterla.

vorrei sottoporre alla sua attenzione una questione che rischia di diventare delicata nella predisposizione del calendario dei lavori parlamentari. Mi riferisco al controverso tema, che campeggia sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, che è oggetto di dibattito e di intervento sia suo sia, con ancora maggiore autorevolezza, per il ruolo, del Capo dello Stato, delle unioni civili. Il Senato ha visto assegnare alla Commissione giustizia i provvedimenti di emanazione parlamentare, e questa è stata una scelta che lei ha fatto e che non mi permetto di sindacare. Intendo sottoporre alla sua attenzione se non voglia,

nei confronti di questo provvedimento. La nostra Costituzione, signor Presidente, prevede una specifica autorizzazione del Presidente della Repubblica quando il Governo presenta disegni di legge in Parlamento. È scritto, infatti, che il Capo dello Stato autorizza la presentazione di disegni di legge. Su una materia come quella al nostro esame, stante la decisione della Presidenza del Senato di assegnare alla Commissione giustizia la discussione dei disegni di legge di natura parlamentare, vorrei capire quali potrebbero essere le sue intenzioni nel caso in cui il Governo, approvato un qualunque disegno di legge, vedesse mancare la sottoscrizione per il concerto

anni addietro. Per l'esattezza nel 1994, anno nel quale fu adottata la legge n. 20 che ridefiniva nel suo complesso l'istituto della responsabilità contabile-amministrativa, e disciplinava in modo specifico l'istituto della prescrizione dell'azione

crisi che investiva le istituzioni, gli apparati pubblici e i partiti politici. Una delle risposte data in quegli anni fu un

ricordiamo che nel 1993 fu adottata la legge sull'elezione diretta dei Sindaci e Presidenti di Provincia. Ebbe inizio un'ampia opera di riforma legislativa tendente a ridefinire gli assetti generali di sistema, in particolare alleggerendo i profili della responsabilità formale, puntando maggiormente sulla capacità sostanziale degli apparati pubblici e delle istituzioni di rispondere

e la responsabilità era integrale, mentre con la legge n. 20 del 1994 si passò ad una prescrizione quinquennale e si espunse la colpa lieve dall'ambito della responsabilità. La legge n. 20 del 1994 puntò quindi a un forte alleggerimento della responsabilità degli amministratori perché, in particolare dal mondo delle autonomie, veniva la domanda di avere un'amministrazione che non dovesse essere assoggettata ad una estrema lunghezza dei giudizi davanti alla Corte dei conti, casi nei quali un amministratore, che magari ormai da 20 anni aveva lasciato il suo incarico, si vedeva assoggettato a giudizio e perseguito per il danno,

importante e rispose ad un intento di sistema. Il quadro normativo è poi rimasto sostanzialmente quello definito con la legge n. 20 (ci fu una leggina un paio di anni dopo, ma per profili minori che non toccano la discussione in quest'Aula). In questo quadro normativo si inserisce il comma 1343

piccola, marginale, ininfluente: dal danno si passa alla condotta produttiva di danno. Invece, anche se apparentemente cambia poco, in termini giuridici cambia moltissimo. Qual è la differenza? È importante cogliere che nella legge del 1994, pur con un alleggerimento del carico quantitativo della responsabilità, si manteneva intatto il modello generale. La responsabilità

e che, per un mio errore di guida (velocità elevata, frenata tardiva, manovra sbagliata), provochi un incidente. Ovviamente la prescrizione per l'azione di danno verso di me decorre dal momento in cui l'incidente si verifica. Supponiamo, invece - secondo esempio che l'incidente si verifichi, non perché ho sbagliato nella manovra, non ho frenato o ho avuto una velocità eccessiva, ma perché anni addietro,

anche in questo secondo caso la prescrizione per il danno da me prodotto decorre dal momento dell'incidente. Diversamente, se si dicesse che quella prescrizione decorre dal momento in cui ho acquistato il pezzo sbagliato e difettoso, che è la condotta produttiva del danno, si potrebbe avere paradossalmente il risultato che il danno è già prescritto nel momento in cui si verifica, perché quel pezzo l'ho acquistato in un tempo antecedente e talmente risalente da aver fatto decorrere l'intero termine di prescrizione prima Ebbene, con il comma 1343 si fa esattamente questo tipo di operazione. In sostanza, il danno dell'amministratore si fa ricadere nella seconda ipotesi. Come se vedessi prescritto il danno da me prodotto guidando l'automobile non dal verificarsi dell'incidente, ma dall'acquisto del pezzo difettoso. Si fa riferimento non al danno che si è prodotto, ma alla condotta produttiva di danno, di danno, che può essere immediatamente antecedente, o anche molto risalente nel tempo. Determinandosi quindi la paradossale conseguenza che potrebbero esservi danni prodotti dall'amministratore già prescritti quanto all'azione di risarcimento nel momento in cui il danno si produce, perché la condotta è precedente di un tempo sufficientemente lungo da aver fatto decorrere il termine della prescrizione.

tengo una condotta: ma temendo che possa venirne un danno, ritardo l'esecuzione fino a quando non mi avvicino talmente al termine di prescrizione da mettermi al riparo dalle possibili conseguenze.

un giusto riconoscimento, di esigenze del tutto ovvie. Tale non è, perché introduce un elemento di grave difformità rispetto al modello generale della responsabilità. Con due ordini di effetti. primo immediato, vale a dire l'effetto sui giudizi in corso con l'azzeramento di un numero che nel momento dell'approvazione della finanziaria non era quantificato è stato possibile quantificare. Ieri in Commissione è pervenuta un'informativa da parte della Corte dei conti che ci ha chiarito che sarebbero molte migliaia i giudizi che verrebbero immediatamente azzerati,

Basti pensare che la condotta produttiva del danno normalmente potrebbe essere la delibera assunta da un organo amministrativo. Ovviamente, fino a quando il danno concretamente si produce non può partire nessuna azione di responsabilità. Magari, il danno si realizza quando si fa un pagamento alcuni anni più tardi, e a quel punto il termine di prescrizione è già

sul transitorio, per intenderci, e uno in termini generali. Evidentemente si tratta di un errore, di uno sbaglio. È chiaro che possiamo porci il problema di velocizzare i giudizi davanti alla Corte dei conti. Ancora adesso sicuramente può capitare e capita che la richiesta di risarcimento venga posta al pubblico amministratore molti anni dopo il verificarsi del danno.

si può e si deve affrontare, ma non agendo sulla prescrizione - questo è il punto - che invece è stato lo strumento utilizzato nella specie. Quindi, non c'è dubbio che questo comma 1343 si dovesse cancellare essendo chiarissimo e indiscutibile l'errore legislativo, fatto con buona intenzione ma con pessimi effetti. Come si poteva cancellare?

Nel dibattito sulla fiducia io stesso ho sottolineato con molta durezza la necessità di porre riparo, e ho argomentato l'inammissibilità

perché vi fosse una valutazione specifica, dal momento che nella pressione dei tempi della mattinata - eravamo nella seduta pomeridiana del 14 dicembre - la Commissione bilancio non aveva colto questo specifico punto.

non diedero il consenso all'apertura di questa «finestra» nella Commissione bilancio. Avendo correttamente il presidente Morando chiesto che vi fosse un consenso unanime dall'Aula, di Forza Italia e AN impedì che si procedesse immediatamente alla soppressione del comma 1343.

Presidente, basta leggere i Resoconti stenografici. Il popolo italiano ci ascolta, i verbali sono su Internet: i cittadini italiani li leggano e vedano chi sono i colleghi che qui, da questo microfono dove io parlo oggi, hanno detto no

a discutere su un singolo comma. Quindi si è scelta la strada del decreto-legge, perché, a quel punto, se non vi era il decreto‑legge il risultato non si poteva conseguire. La finanziaria produce effetti dal 1° gennaio. Una legge ordinaria sarebbe comunque entrata in vigore dopo e quindi, siccome la prescrizione è una fattispecie a effetto istantaneo, comunque si sarebbe avuto l'effetto estintivo e si sarebbe poi dovuto intervenire retroattivamente su una fattispecie estinta con una grave rottura dei principi. Invece era possibile, essendo la finanziaria promulgata e pubblicata ed essendo la finanziaria stessa una legge a effetto differito, perché gli effetti si producono dal primo gennaio, nell'intertempo tra la promulgazione e la pubblicazione e il prodursi degli effetti si poteva intervenire con un decreto che cancellasse la norma. A questo punto è sorta una questione: si può o non si può intervenire dopo la promulgazione e pubblicazione e prima, nel caso della finanziaria, del primo gennaio? Esiste, cioè, la norma in quell'intertempo? Perché è questa la domanda dal punto di vista giuridico. Non vi è dubbio che esista. La promulgazione e la pubblicazione servono esattamente a far entrare la norma, secondo quello che dicono i manuali, nel sistema giuridico e, come tale, da quel momento la norma Che poi produca i suoi effetti o no è altra questione: può produrli dopo, molto dopo, poco dopo, subito, ma questa è una cosa che può essere diversamente disciplinata dalla stessa legge. Non vi è dubbio che, nel momento della promulgazione e della pubblicazione, viene in esistenza la norma giuridica, che quindi diventa oggetto di un possibile intervento da parte di successiva norma.

Supponiamo che la legge "B" non venga mai adottata. Secondo la mia tesi posso avere una legge "C" che vada ad abrogare la legge "A", e la cancelli dal sistema giuridico. Secondo la tesi contrapposta, che oggi nega la possibilità che il decreto tocchi il comma 1343 della finanziaria, una legge "C" non potrebbe mai cancellare la legge "A", che rimarrebbe indefinitamente agli atti, pur non producendo mai alcun effetto.

1343 da una successiva legislazione, prima del 1° gennaio e, quindi, del prodursi dei suoi effetti. Naturalmente, è vero che il decreto-legge poteva anche teoricamente avere un contenuto diverso:

Ma a quel punto la scelta politica opportuna era quella di abrogare, e non già di operare in modo diverso sul comma 1343. Dunque, il decreto era tecnicamente possibile, doveroso e politicamente opportuno, perché era stato fatto un errore, perché con il comma 1343 era stato preso un indirizzo sbagliato, soprattutto in un momento in cui - esprimo la mia personale opinione su questo - non si avverte l'utilità o il bisogno di ulteriori alleggerimenti della responsabilità degli amministratori. Anzi, forse bisogna pensare ad un rafforzamento delle tutele giuridiche della buona e corretta amministrazione, perché si sono indeboliti i meccanismi della responsabilità politica e istituzionale, soprattutto nel mondo delle autonomie (come ho detto già nel dibattito sulla fiducia),

conclusione. Con le mie considerazioni non intendo affatto censurare i colleghi che hanno opinioni diverse dalle mie e che hanno presentato e sostenuto l'emendamento. Più volte nel corso degli anni è stato fatto il tentativo di alleggerire le forme giuridiche della responsabilità degli amministratori. Anche io ho ricevuto in più occasioni non ho mai accettato. Tuttavia credo che ogni parlamentare risponda alle sollecitazioni secondo la sua esperienza, i suoi mondi di riferimento,

tutte le istanze e le sollecitazioni. Quindi, ribadisco che non censuro in nessun modo i colleghi che si sono fatti portatori e sostenitori di questa istanza, anche se, come ho detto, non la condivido.

ripreso nel maxiemendamento governativo, nonostante che - come emendamento - fosse stato esplicitamente respinto dalle forze politiche della maggioranza. Perché anche questo va detto. Noi non dovremmo trovarci qui a discutere oggi di questo decreto. Si dice sia stato un errore. Forse. Ma rimane un punto politico rilevante, che attiene al corretto rapporto tra l'istituzione Parlamento e l'istituzione Governo, chiunque governi e chiunque sia opposizione. Il punto è che il Governo non deve mancare agli impegni assunti con la propria maggioranza. Invece, questo è accaduto con il comma 1343 e con altri punti - non pochi - della legge finanziaria. Voglio dirlo pacatamente, ma con fermezza, perché dimostra innanzitutto che non si può rozzamente disegnare sulle istituzioni un copione in cui i cattivi sono in Parlamento e i buoni sono al Governo. Non è così.

Il decreto-legge consiste nella pura e semplice abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, al fine di correggere quello che il Governo definisce nella relazione al disegno di legge di conversione un "mero errore redazionale". Alla luce dei criteri particolarmente rigorosi cui la Presidenza deve attenersi sulla base della prassi conseguente alla pronuncia della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984, in relazione ad emendamenti presentati a decreti-legge, risultano proponibili gli emendamenti 1.0.107, 1.0.108 e 1.0.109, del senatore Castelli, nonché 1.101 e 1.102, del senatore Storace. Sono invece improponibili, per estraneità all'oggetto, gli emendamenti 1.0.1, del senatore Martinat, 1.0.101, 1.0.102 e 1.0.103, del senatore Saporito, e 1.0.104, 1.0.105 e 1.0.106, del senatore Salvi, in quanto tendono a modificare commi diversi della legge finanziaria 2007 o del decreto-legge collegato. perché privi di portata normativa, gli emendamenti 1.1, del senatore Carrara, e 2.100 e 2.101, del senatore Castelli. Sono inoltre improponibili gli emendamenti 1.103, avente il contenuto tipico di un atto di indirizzo al Governo, 1.104, perché incide sull'esercizio di diritti individuali non comprimibili con legge ordinaria,

Signor Presidente, come sempre mi rimetto scrupolosamente alle decisioni della Presidenza. Lo faccio anche in questa occasione. Mi permetta di esprimere l'auspicio che un criterio così rigoroso sia applicato dalla Presidenza in tutta la prossima fase della legislatura. Si discute molto di legge finanziaria e di una sua eventuale riforma. L'argomento oggi all'esame dell'Aula è legato certamente ad una vicenda che il Presidente della Repubblica ebbe a definire una mostruosità giuridica in occasione di un suo intervento. Ebbene, è mio convincimento, signor Presidente, che premesse tutte le possibili, opportune norme legislative e modifiche regolamentari che si ritenga di introdurre, vi sono già oggi alcune regole, come per esempio il divieto di introdurre in finanziaria (e presumo si debba ritenere anche negli emendamenti o nei maxiemendamenti alla legge finanziaria) norme ordinamentali e microsettoriali. Essendo tale scrutinio affidato ai Presidenti delle Assemblee, ritengo che l'indirizzo intrapreso oggi sia di buon auspicio perché nelle prossime leggi finanziarie il potere di controllo dei Presidenti delle Assemblee sia usato con estremo scrupolo e rigore anche per i futuri provvedimenti che saranno al nostro esame, onde evitare - come ci è accaduto - di votare in blocco anche al di fuori della finanziaria provvedimenti legislativi. Mi riferisco in particolare a due decreti-legge, nei quali inopinatamente erano inserite norme o di *spoils system* o di analoghe caratteristiche come il tema di finanziamento dei partiti, del tutto estranee a questa materia e che pongono i parlamentari della maggioranza nella difficile condizione se dover dire sì o no in blocco ad un provvedimento che condividono in buona parte ma di cui non accettano singoli punti, introdotti senza che vi siano stati dibattito e confronto parlamentare. Nell'accettare quindi questa sua decisione, esprimo l'auspicio che analogo rigore sia seguito in futuro nei confronti di emendamenti, siano essi presentati dai parlamentari sia dal Governo. finestra"). Consapevolmente sottolineo il suo rilievo perché questo precedente resti come punto di orientamento anche per il futuro.

che possono derivare dall'attuazione del comma 1343 e riteniamo del tutto inidoneo lo strumento utilizzato dal Governo con il decreto-legge, per le ragioni che magari verranno rese in termini più chiari in dichiarazione di voto, ma che sostanzialmente si incentrano sulla possibilità o meno di abrogare una norma che ancora non è entrata in vigore.

e, consapevoli che nel procedimento legislativo alla fase del varo in copia conforme da parte della seconda Camera del Parlamento, quindi alla fase della perfezione della legge, consegue quella della pubblicazione e della vigenza, riteniamo che il legislatore possa intervenire correttamente su una legge perfetta, ma non ancora vigente. Ebbene, qual è il punto? Invece di abrogare una

in vigore, invece di perseguire un'operazione che per essere legittima sotto il profilo del procedimento legislativo richiede la vigenza della legge abrogata sia pure per un secondo come l'applicazione, ove possibile, del principio del *favor rei*, di cui all'articolo 27 della Costituzione, si poteva tranquillamente operare sul testo del comma 1343 e quindi condizionare la sua entrata in vigore ad una previa modifica; il che evidentemente avrebbe impedito la vigenza, sia pure per un secondo, del comma 1343. Presidente, se non ho capito male, l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che tale comma sarebbe privo di portata normativa, raggiungerebbe cioè gli stessi effetti abrogativi di cui al decreto-legge. Mi permetto, signor Presidente, di rappresentare che a mio avviso ciò non è. Infatti, mentre il decreto‑legge, parlando di abrogazione, richiede, secondo dottrina, dottrina, l'entrata in vigore della legge abrogata, sia pure per un secondo, questo comma impedisce l'entrata in vigore di quella legge sia pur per quel secondo, e quella vigenza di un secondo potrebbe essere foriera di conseguenze non piacevoli e gravemente dannose sotto il profilo economico del nostro Paese. Vorrei fare un ultimo rilievo, signor Presidente, evidentemente prendendo atto della sua decisione. Nelle discussioni che si sono svolte in Commissione si era proposta una riformulazione dell'emendamento, nel senso

la modifica. Solo questo dimostra, essendosi ritenuto possibile intervenire su una legge perfetta ma non ancora vigente toccando la data di vigenza, la possibilità di intervenire su una legge perfetta, quindi di andare a modificare il testo. Personalmente, Presidente, le segnalo che a mio modestissimo avviso tale soluzione sarebbe per certi versi più idonea e sicuramente più tranquillizzante rispetto a quella contenuta nel decreto-legge. Mi permetto di farle osservare, signor Presidente, che a mio avviso vi è portata normativa, perché l'emendamento comunque impedirebbe l'entrata in vigore del comma che si vuole abrogare,

un atto che francamente, secondo me, è davvero sbagliato, perché si vuole impedire al Senato di misurare la portata di una norma proposta e credo ciò sia grave. Anzitutto, contesto, Presidente

avrebbe potuto far svolgere tranquillamente la discussione generale, verificare gli orientamenti dei Gruppi sul tema oggetto della nostra discussione e poi determinare l'Assemblea, attraverso gli orientamenti che ella avesse voluto dare, alla discussione degli emendamenti. Lei ha preferito la strada inversa per strozzare il dibattito e ciò non va bene. In secondo luogo, è abbastanza imbarazzante leggere questa nota, perché fa riferimento ad una pronuncia della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984. Ora, Presidente, abbia almeno la cortesia di fornire ora per il futuro questa benedetta delibera, perché è impensabile che il Senato, Senato, quando presenta gli emendamenti, debba svolgere un minuzioso lavoro di ricerca risalente addirittura all'8 novembre 1984, perché non si può parlare di queste norme. Non credo sia corretto agire così nei confronti del Senato, soprattutto quando siamo in presenza di un numero limitatissimo di emendamenti. La terza questione che le propongo è la seguente. Lei fa bene a dare atto al presidente Salvi della necessità di affermare un precedente per il futuro, ma guardi, Presidente, la tesi per la quale sostanzialmente si ricorre a una sorta di estraneità di materia si evince da alcune delle affermazioni contenute in questa nota. Ma lei l'ha letta la legge finanziaria che ha fatto passare qui, il maxiemendamento del Governo? Vogliamo capire se, in base a questa norma decisa dalla Giunta per il Regolamento nel novembre del

francamente trovo assolutamente ingiustificata la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.103. Proprio la legge finanziaria, presidente Marini,

nuova finestra"). Per quanto riguarda lo strozzamento del dibattito, c'è tutta la discussione generale alla quale lei ha fatto riferimento a conclusione del suo intervento.

accetti l'invito a non intervenire nei confronti della stampa da parte dei singoli. Come emendamento, come decisione legislativa mi pare assolutamente impropria. Naturalmente ci sono altri strumenti che possono essere utilizzati. Queste sono le motivazioni. Del resto,

dei dirigenti. Signor Presidente,rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, nessuno si aspetti che intervenga per fatto personale. Chi dovesse pensarlo commetterebbe un grave errore, pur essendo vero che da più di un mese verso di me e contro di me sono state sprecate qualificazioni estremamente spiacevoli, ai limiti della diffamazione, che, partendo da una lettura estremamente superficiale di quanto sto per rappresentarvi, sono arrivate a valutazioni tanto ridicole quanto infondate. Poiché tali considerazioni sono il frutto di una totale disinformazione, spero colposa e non dolosa, formulata sulla base di dati fattuali inesistenti e tendenziosi, la *ratio* del mio intervento è quella di fare finalmente un po' di chiarezza sui punti fondamentali di un emendamento normativo, che è stato oggetto di tante critiche infondate ma di nessun approfondimento. Il comma 1343 del maxiemendamento alla finanziaria, quel comma della discordia, che per lungo tempo molti hanno impropriamente battezzato con il mio nome, è stato estrapolato, con modalità alle quali sono del tutto estraneo, dal testo di un emendamento ben differente dall'interpretazione altrettanto impropriamente veicolata nelle ultime settimane. L'emendamento originario, di cui rivendico - di quello sì - la più completa e totale paternità, era un testo ben diverso, completo ed articolato, che nel pieno rispetto del termine quinquennale di prescrizione, rimasto fermo ed immutato, rispondeva e risponde ad un'istanza di civiltà giuridica. Nella sua formulazione, l'emendamento aveva due obiettivi fondamentali: da una parte, mirava a dare effettività al termine quinquennale, rendendolo non suscettibile di interpretazioni abnormi, che in concreto l'hanno fatto diventare ultradecennale; dall'altra, voleva ribadire il principio della personalità della responsabilità e conseguentemente dell'illecito dell'amministratore e del pubblico dipendente, affermato dall'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, in attuazione dell'articolo 28 della Costituzione. E ciò in aderenza a due principi fondamentali, il primo in materia di responsabilità, ove è incontroverso che il termine prescrizionale decorre di regola dalla commissione dell'illecito; il secondo di rilevanza non solo costituzionale ma anche comunitaria, della ragionevole durata del processo, in tutti i procedimenti in cui esso si articola, principio questo impostoci anche dall'articolo 6 del Trattato di Roma del 1950, che ha sancito la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e in materia la cosiddetta legge Pinto insegna. Nelle ipotesi di danno indiretto, che costituiscono l'oggetto specifico dell'emendamento in argomento, non può considerarsi ragionevole che il termine prescrizionale si ampli a dismisura per decenni e decenni dal compimento della condotta ritenuta produttiva di danno erariale, esponendo l'indagato *sine die* anche all'incubo di un procedimento sanzionatorio la cui conclusione può portare alla rovina economica oltre che morale del soggetto stesso e della sua famiglia. In tale contesto intendo evidenziare ancora una volta che il problema esiste, è reale e va affrontato con urgenza, per cui si sarebbe potuto discutere non dell'oggetto di intervento normativo, bensì semmai della formulazione, sempre perfettibile, e dell'organicità e della completezza della norma invece di continuare a disinformare e a cercare lo scandalo dove non c'è. Basterebbe una domanda per comprendere l'abnormità della tesi portata avanti in quest'ultimo mese e di cui ancora oggi non riesco a comprendere le ragioni: come si può ammettere che, fermo restando il principio legale secondo cui la prescrizione è quinquennale, alcuni soggetti (dirigenti ed amministratori) in via di interpretazione in via di interpretazione possano essere perseguiti dopo decenni e decenni, in via indefinita o addirittura *sine die*; e come è accettabile, agendo dopo decenni, continuare a denominare quinquennale la prescrizione senza cogliere l'abnormità di una simile situazione? appunto, e solo questa, si voleva eliminare, imponendo che l'azione venga intrapresa comunque entro i cinque anni dal verificarsi della condotta imputata al pubblico amministratore e consentendo a quest'ultimo la possibilità concreta di difesa quale garanzia del giusto processo. E ciò, lo si sottolinea, senza alcun pregiudizio per l'azione dell'autorità inquirente, neppure sotto il profilo del carico di lavoro da svolgere nel termine di legge, posto che nei cinque anni è sufficiente per scongiurare la prescrizione la semplice immissione di un atto interruttivo e sempre considerando che per il danno indiretto il procedimento può essere sospeso fino alla definizione del giudizio, come peraltro espressamente previsto dal comma 2 dell'emendamento da me presentato. La mia proposta, in particolare, era rilevante ed applicabile non a tutti i giudizi, ma essenzialmente alle tipologie per danno indiretto caratterizzato dalla responsabilità per danni causata a terzi liquidati a seguito di giudizio civile da essi proposto contro l'amministrazione. Solo per il danno indiretto, infatti, vi può essere una sensibile divergenza tra la data dell'illecito e quella di produzione del danno maturato a seguito di un giudizio autonomo. Il caso più ricorrente, che rappresenta la quasi totalità dei processi già avviati o che potranno ancora essere avviati, è quello della convocazione in giudizio per responsabilità discendente dalla mancata definizione dei termini di procedura espropriativa, divenuta irregolare e perciò causa di azione di risarcimento da parte del proprietario. Il giudizio civile risarcitorio intentato dai proprietari lesi contro l'amministrazione espropriante si conclude al termine dei lunghissimi tre gradi previsti, con l'ovvia ed assurda conseguenza che le cause si perpetuano per decenni. In tali ipotesi l'indagato, amministratore o pubblico dipendente, che sia chiamato a rispondere davanti alla Corte dei conti dopo tanti anni si trova nell'impossibilità concreta di difendersi, non avendo più la disponibilità o la reperibilità di atti, documenti o posizioni amministrative legittimanti. Infatti il pregiudizio irreparabile è accresciuto ulteriormente proprio dalla circostanza che egli non ha avuto la possibilità di intervenire nel giudizio dal cui esito discende il danno erariale che è chiamato a risarcire; e quando un cittadino è accusato e condotto in giudizio senza alcuna possibilità concreta ed attuale di difendersi, dopo essere stato depauperato degli elementi utili alle sue argomentazioni, visto il lungo tempo trascorso, si verifica quanto ottimamente evidenziato dal dottor Pelino Santoro, illustre giurista e presidente di sezione della Corte dei conti, che ha scritto (leggo testualmente): «Non c'è giudice che, se pur gli darà in definitiva ragione, possa cancellare il senso dell'ingiustizia subita e da lui avvertita come un sopruso, un affronto, un'ignominia, spesso irreparabile quanto meno per occasioni perdute e l'onore offuscato». Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo si possa negare il macroscopico danno, che ha il sapore di una beffa, cui il mio emendamento voleva porre rimedio, anche per impedire la violazione del fondamentale diritto alla difesa garantito costituzionalmente. Ed invece si è parlato di «colpo di spugna» per «reati contabili», di pericolo di prescrizione per quasi 70.000 processi, di famigerato intervento atto ad agevolare dei delinquenti, tanto per ricordare alcune tra le affermazioni più ricorrenti; affermazioni, però, tanto immotivate quanto non rispondenti alla realtà né alla verità, come sarebbe stato agevolmente accertabile con una semplice verifica fattuale, al lume dei più elementari principi di diritto.

né una riduzione del termine prescrizionale che era e resta quello di 5 anni stabilito dalla legge n. 20 del 1994 che, a sua volta, aveva ridotto il termine ritenuto decennale dalla giurisprudenza previgente. La mia proposta voleva invece rendere effettivo il termine stesso, non consentendo che, con l'applicazione di una semplice e tendenziosa interpretazione, si potesse continuare a portarlo oltre i 20 anni, se non *sine die*, spostando artificiosamente, per alcune tipologie, il termine iniziale, cosicché in tal modo il quinquennio non comincerebbe mai a decorrere. Fermo restando l'istituto della prescrizione quinquennale, l'emendamento si riferisce ‑ e ciò si è volutamente ignorato - non a tutti i procedimenti davanti alla Corte dei conti ma solo ed esclusivamente a quelli concernenti i casi già richiamati di responsabilità per danni indiretti che - ripeto - non sono conseguenza immediata degli atti illegittimi, perché richiedono come presupposto l'espletamento di un altro giudizio alla fine del quale si produce il danno. L'emendamento non si riferisce nemmeno lontanamente ai danni diretti in cui il comportamento illegittimo provoca direttamente ed immediatamente l'evento dannoso, e dunque non vi può essere un rilevante stacco temporale tra la condotta illecita sanzionabile ed il danno prodotto dalla condotta medesima: in tali casi il danno è conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, pertanto la prescrizione si prevede sempre a decorrere da tale data, che è comune alla conclusione dell'illecito ed alla produzione del danno. Se si escludono - come devono essere esclusi - i danni diretti, l'oggetto di tanta discordia, anche dal punto di vista dei dati statistici, si riduce a ben poca cosa, come vedremo tra poco. Ma prima, ancora più incisivamente, è indispensabile negare nel modo più categorico ed assoluto il pericolo di prescrizione per effetto della norma in esame, poiché la normativa non potrebbe mai essere applicata ai casi ed ai processi pendenti e preesistenti. È infatti noto a tutti che, di regola, la legge opera solo per l'avvenire e che la retroattività deve essere espressamente disposta, salva la tutela dei diritti acquisiti. Pertanto, in nessun caso - lo ripeto con forza - potrebbe ipotizzarsi l'applicazione retroattiva della norma concernente la prescrizionale. Per eliminare in radice anche solo la possibilità di una discussione in merito, il caso ha voluto che la questione di diritto sia stata già affrontata e risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza della stessa Corte dei conti. Tale precedente è stato fissato quando, a seguito della legge n. 20 del 1994, il termine prescrizionale, nei giudizi davanti alla Corte dei conti, è stato ridotto da 10 a 5 anni. In tale occasione dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto pacificamente che ai procedimenti pendenti si continuasse ad applicare il precedente termine decennale, come è agevole verificare dalla semplice lettura del classico manuale sui «Giudizi innanzi alla Corte dei conti» di Francesco Garri, già procuratore generale della stessa Corte, in cui è detto che il più breve termine prescrizionale «si applica ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della norma che lo prevede», per cui ai fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del nuovo termine continua ad applicarsi la normativa pregressa, sulla scorta della ivi richiamata pacifica giurisprudenza anche delle sezioni riunite della Corte dei conti nonché della Corte costituzionale. È infine appena il caso di specificare che, per argomentare sulla retroattività della legge civile ed amministrativa, non ha rilevanza (ed è del tutto fuori tema) il principio di diritto, applicabile solo alla legge penale (ed espresso dall'articolo 2, comma 2, del codice penale), secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la posteriore sono diverse, si «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo». Tale norma è propria, infatti, solo ed esclusivamente della legge penale (ed è correlata all'articolo 25, comma 2, della Costituzione) e si riferisce a «reato» e «reo», non ad altre figure giuridiche soggettive. Deve essere chiara e indiscutibile, dunque, l'impossibilità assoluta di sostenere che la norma amministrativa successiva avrebbe potuto essere applicata retroattivamente in quanto più favorevole, poiché l'estensione della norma penale al procedimento amministrativo costituirebbe un plateale «errore di grammatica», smentito anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha sancito l'irretroattività nell'identica fattispecie di successione di leggi relative alla prescrizione per la Corte dei conti, escludendo, ovviamente, la possibilità di ipotizzare l'applicabilità di altro principio. Ancora più grave è stato il lasciar intendere surrettiziamente che si potrebbero prescrivere i processi già iniziati, il che non può essere affermato in buona fede: tutti sanno, infatti, che, mentre nel diritto penale per i reati sono previsti termini massimi entro cui il procedimento deve essere concluso per non incorrere nella prescrizione, nel giudizio dinnanzi alla Corte dei conti è sufficiente che nei 5 anni si dia inizio al procedimento, anche con un semplice atto interruttivo, che può essere l'invito a dedurre o una richiesta scritta. Nella sostanza, poi, tutto l'allarme ed il clamore cui abbiamo assistito discendono da un dato di fatto iniziale, recepito dagli organi di stampa nella sua totalità, che è tanto suggestivo quanto falso: quello secondo cui l'emendamento opererebbe «un colpo di spugna» per quasi 70.000 processi, con effetti devastanti sull'erario, con specifico riferimento alle frodi comunitarie. Niente di più falso, colleghi senatori, perché l'ammontare di circa 70.000 processi (per l'esattezza 68.760) concerne l'intero contenzioso e, cioè, tutti - e dico tutti - i processi pendenti davanti alla Corte dei conti ed in tutto il territorio nazionale, di cui i casi di illeciti contabili per danni indiretti rappresentano una porzione più che esigua. Per la maggior parte dei 70.000 processi, fondamentalmente relativi a danni diretti, l'emendamento non potrebbe avere, quindi, alcun effetto, anche indipendentemente dalla non retroattività. Tanto meno potrebbe avere effetto per le tipologie specificamente indicate come le più rilevanti (consulenze illegittime, erogazioni illecite di fondi comunitari, trattamento del personale), per le quali, anche solo facendo uso del buon senso, chiunque è in grado di comprendere che il danno è contestuale al comportamento illegittimo che ha effettuato le spese illecite, per cui non ha alcuna conseguenza l'emendamento che fa decorrere la prescrizione dal verificarsi dell'atto illecito. Per i medesimi motivi l'allarmistico e tendenzioso dato eccepito, secondo cui vi sarebbe stato il rischio di prescrizione, con una perdita di 310 milioni di euro solo per le frodi comunitarie, è completamente fuori della realtà, perché, sempre a prescindere dall'irretroattività della norma, si tratta comunque di danno diretto, immediatamente perseguibile. È poi incredibile che chi ha affermato di preoccuparsi di tale pericolo, completamente irreale, non abbia ricordato che, trattandosi di reati, è applicabile la normativa sulla prescrizione penale. E per i reati produttivi di danno il risarcimento viene comminato normalmente dal giudice penale, a seguito di costituzione di parte civile, doverosa per l'amministrazione. Nessuna prescrizione, dunque. Nessun colpo di spugna nell'intento di premiare gli amministratori passibili di illegittimità. Anzi, ritengo necessario puntualizzare che l'originario emendamento da me proposto, lungi dal giustificare un intento lassista, conteneva disposizioni che inasprivano l'attività di rilevamento e di sanzione degli illeciti contabili, come facilmente verificabile. Onorevoli colleghi, in tale contesto ben si comprende che la norma non solo non provoca alcun danno, anche in relazione al suo ristretto ambito di applicazione ed alla sua irretroattività, ma è anzi espressione di civiltà giuridica ed applicazione di principi di rilevanza costituzionale e comunitaria. L'unico pericolo, semmai, potrebbe discendere dalla mancata regolamentazione, secondo giustizia, della materia. Occorre procedere, senza perdere tempo, alla formazione di una legge giusta, non per proteggere chicchessia, ma per porre fine all'indeterminatezza della durata dei processi e per garantire l'inviolabile diritto alla difesa. Ricordando anche che, quando più di qualcuno si è accanito, inspiegabilmente, nel tentativo di affermare responsabilità amministrative dei politici, ha fatto opera retrospettiva e di retroguardia: ora, dopo la fondamentale riforma che ha sancito la scissione tra la competenza degli amministratori per gli atti politici e di indirizzo e quella dei dirigenti per gli atti di gestione, non è più ipotizzabile, per la generalità dei casi, una responsabilità contabile degli amministratori, poiché la responsabilità medesima consegue ad atti di gestione di competenza dei dirigenti. Signor Presidente,rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, concludo affermando che il legislatore ha forte l'obbligo di rivedere l'intero istituto dell'azione di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti, con specifico riferimento al problema dibattuto della durata e della data di decorrenza della prescrizione. Sono certo di aver portato all'ordine del giorno del legislatore un argomento ed una proposta sani ed opportuni, per tutte le ragioni che ho appena illustrato, e confido nel riconoscimento della fondatezza e giustezza di quanto ho esposto. Oggi, il decreto di cui stiamo trattando viene definito come atto opportuno, in quanto si ritiene non conveniente che una legge finanziaria contenga disposizioni di carattere ordinamentale e perché, come si legge nella relazione che lo accompagna, l'inserimento di tale norma nell'ambito della legge finanziaria 2007 è risultato il frutto di un mero errore redazionale. Mi permetterete, in chiusura, di ricordare e sottolineare, affinché sia chiaro e indiscutibile per tutti, che non ho nulla a che vedere con la stesura del maxiemendamento e che nello specifico, il fantomatico comma, di cui stiamo dibattendo la ratifica della cancellazione, è attinente ad un errore redazionale che non mi concerne e che nemmeno conosco. STORACE smembrando la mia proposta di emendamento e privandola dei suoi elementi caratterizzanti e rilevanti, ha dato il via ad una serie di fuorvianti interpretazioni ed ha leso non solo il testo da me presentato, ma soprattutto la possibilità di comprendere un argomento importante ed urgente come quello di cui stiamo discutendo. Al Governo e a questo Senato, che sono sicuro condividono l'importanza e la serietà dell'istituto o dell'azione di responsabilità contabile, chiedo un impegno diretto a legiferare, e subito, rivisitando la materia e ristabilendo con chiarezza definitiva il *dies a quo* della decorrenza del termine quinquennale della prescrizione. Fiducioso che ciò avvenga, voterò il decreto.

e morta all'interno dell'attuale maggioranza di centro-sinistra. Non c'entra assolutamente l'opposizione su questa vicenda. Avete fatto tutto voi. E credo sia giusto ricostruire, sia pure brevemente,

probabilmente quella di chiudere con un numero consistente di procedimenti pendenti presso la Corte dei conti, però poi è stato il dibattito all'interno del centro-sinistra che ha

rispetto al precedente Governo di centro-sinistra. Cercheremo e colpiremo fino in fondo i responsabili dell'inserimento di questa norma nella legge finanziaria». Ebbene, ieri innanzitutto il Governo è venuto spiegarci chi è stato il responsabile dell'inserimento di questa norma nella legge finanziaria. Sapete chi è stato? È stato il computer! Non Non è stato un uomo, un rappresentante del Governo o un alto funzionario dello Stato, bensì il computer che, avendo avuto disposizione di cancellare tutti i commi all'interno della finanziaria in cui risultavano le parole

che, come ha già spiegato, aveva un altro obiettivo, cioè di affrontare una volta per tutte la vicenda del danno indiretto. Non è possibile che in Italia,

Chiaramente siamo stati richiamati dall'Alta Corte europea per la durata dei processi che non ha pari nel genere in tutta Europa. Ritengo che sicuramente il responsabile non sia stato il

Il numero dei giudizi fatalmente destinati all'estinzione e l'ammontare del complessivo netto delle condanne», che sarebbero travolte dalla mancata conversione

e le condanne già espresse in primo grado sono pari a 814 milioni di euro, a cui si devono aggiungere le rivalutazioni monetarie, gli interessi legali e le spese di giustizia, con un'incidenza che, alla fine, porterebbe la cifra ad alcuni miliardi di euro». Dunque, dietro questo emendamento una valutazione estremamente consistente in termini economici. dice sempre il procuratore generale della Corte dei conti: «Vi è il rischio che la norma in questione vanifichi il recupero di ingenti importi, quali i 32 milioni di euro recentemente versati in esecuzione di un'unica condanna al Comune di Roma». L'unico caso che viene citato è una vicenda relativa al Comune di Roma. Allora mi chiedo: è possibile che sia stato il computer ad inserire questa norma?

che sono coinvolti in questi procedimenti che rischiavano di essere estinti e credo che ne vedremmo delle belle. Io credo che vedremmo, all'interno di questo elenco, nomi molto noti della politica e dell'amministrazione italiana, e sarebbe una cosa importante che per ragioni di trasparenza questi nominativi venissero resi pubblici. Ho voluto dire queste cose perché immagino a parti invertite, se fosse stato all'opposizione il centro-sinistra, voi, come avete fatto nella passata legislatura, avreste bloccato il Parlamento, organizzato girotondi, gridato ai colpi di spugna, avreste, in sostanza, mobilitato la piazza contro un provvedimento di questo genere. Se invece lo fate voi, viene ridotto a semplice errore materiale provocato da un computer. Io credo che questa spiegazione Nello stesso tempo, però, devo dire che le questioni poste dal senatore Fuda vanno affrontate con un disegno di legge, autonomo evidentemente, non all'interno di questo provvedimento. Si deve ragionare in modo equilibrato su come ridurre i tempi decennali per arrivare a un giudizio da parte della magistratura contabile. Non possiamo tenere migliaia di amministratori e di funzionari *sub iudice* e rovinargli la vita: le colpe vanno affrontate, i danni vanno definiti nei tempi più brevi possibili, non certo in vent'anni, e il senatore Fuda ha completamente ragione. Da parte nostra daremo tutta la collaborazione possibile un'intesa su un provvedimento che risolva le questioni sul danno indiretto poste dal senatore Fuda. Concludendo, signor Presidente signor rappresentante del Governo, questa è una vicenda che non va trasformata, come cercate di fare voi, in mero errore tecnico, edulcorata, difesa e coperta ipocritamente. La mia convinzione è che talvolta a pensare male si pensa bene, come diceva e dice spesso il senatore Andreotti. Sono convinto che la manina che ha inserito questa norma aveva un ben chiaro disegno ed è quello che vi ho detto. Quando si conosceranno i 3.400 nomi che sono sottoposti a procedimento da parte della Corte dei conti già in primo grado ne vedremo delle belle e sarebbe bene, per finirla in questo Paese in cui tutti fanno i giustizialisti - io faccio parte di un'altra cultura e di un altro mondo che si rendessero pubbliche queste informazioni, così si farebbe chiarezza in questo Paese che talvolta veramente sposa solo posizioni populiste e giustizialiste che stanno facendo un male profondo a tutta l'intera nostra comunità.

la questione, come è stato già richiamato dal relatore e da alcuni interventi, è in discussione perché è stato commesso un errore. Vorrei citare il collega senatore a vita che dice che a pensare male si va vicino alla verità, ma non credo che la Corte dei conti potrà rifarsi su Bill Gates per eventuali danni. Penso sia utile ragionare, al di là dei richiami che il senatore Villone faceva ad atteggiamenti assunti dalle varie rappresentanze politiche, sul da farsi, sulle opportunità: a questo punto della situazione, allo stato dell'arte, qual è l'atteggiamento da assumere, la scelta che consenta di mantenere ancoraggio alla giustizia, alla dignità delle persone e anche all'impressione che abbiamo lasciato, che non è stata certo bella. La stampa si è sbizzarrita ad individuare possibili beneficiari di questo errore materiale. Penso che per tutti valga il principio della presunzione di innocenza, ritengo tuttavia che il provvedimento oggi al nostro esame sia la soluzione migliore che abbiamo di fronte, nonostante la discussione in punta di giurisprudenza o di competenza costituzionale che suggeriva l'adozione di un provvedimento che facesse slittare i tempi, dando così modo e tempo per l'adozione di un provvedimento legislativo. si tratterebbe comunque di intervenire con una modifica di quanto disposto dalla legge finanziaria; quindi, ragionevolmente, con buon senso, ma anche sulla base degli esempi del passato che sono stati richiamati quanto ad applicazioni, credo sia opportuno adottare questo decreto.

abbiamo determinato un alleggerimento di responsabilità da parte degli amministratori e un aumento di responsabilità da parte dei tecnici.

agli amministratori e, ancor più, all'opinione pubblica la possibilità di partecipare alle scelte fatte da un ente locale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'abrogazione del comma 1343 della finanziaria 2007, lì inserito nelle ultime, convulse ore che hanno preceduto la sua redazione finale, è un atto doveroso da parte del Parlamento, che in questo senso si era già espresso durante la discussione in Aula sulla stessa finanziaria, ma che non aveva potuto procedere allora alla sua cassazione perché alcune forze di minoranza avevano fatto mancare quella unanimità necessaria ad intervenire in quella delicata sede. Oggi quindi rimediamo ad un errore, ma non saremmo onesti con noi stessi se non riconoscessimo il caso del comma 1343 ci rimanda ad almeno tre altre questioni rilevanti che qui, per brevità di tempo, semplicemente richiamiamo con i titoli, ma che il Parlamento dovrà affrontare e risolvere in modi e tempi certi. Esse sono, appunto, i tempi della giustizia, la certezza del diritto e la formazione della legge di bilancio. Sui primi due aspetti condividiamo, nella parte analitica, la relazione del senatore Villone, la quale allude, ci sembra, alla necessità di una verifica proprio sui tempi e i modi che garantiscono l'erario, da una parte, e gli amministratori, dall'altra. Sulla legge di bilancio vi è un ampio consenso affinché si arrivi ad una sua riforma. Già nei prossimi giorni le Commissioni bilancio della Camera e del Senato inizieranno un percorso di studio, comprensivo di audizioni, per offrire al Parlamento una o più proposte su cui confrontarci. È necessario, tra l'altro, in riferimento allo stesso comma 1343, restituire la massima trasparenza e capacità critica e decisionale al Parlamento, il quale - è questa la nostra sensazione - nell'ultima finanziaria si è trovato di fronte ad alcune decisioni e scelte che non hanno avuto a che fare con un confronto democratico corretto. Il collega Fuda ha ricordato come l'emendamento da lui firmato, ma sottoscritto da altri colleghi, nell'originale constava di tre commi, effettivamente più bilanciati nel loro insieme dell'unico sopravvissuto nel comma 1343. Nessuno finora ha potuto stabilire una versione condivisa di come si sia giunti a questo risultato. Noi, per parte nostra, abbiamo raccontato la vicenda sul nostro quotidiano di Rifondazione, "Liberazione", per come l'abbiamo potuta ricostruire. Di certo, appare chiaro che la decisione finale è stata sottratta sia alla Commissione bilancio sia all'Aula. Quindi, anche per evitare che posizioni tecniche finiscano col prevalere sulla decisione politica, annunciamo fin da ora il nostro massimo impegno affinché si possa approvare, speriamo entro l'estate, quindi al più presto, una riforma della sessione di bilancio. Con queste motivazioni, voteremo favorevolmente alla conversione del decreto-legge in

perché ritengo irrispettoso da parte del Governo venire nelle Aule parlamentari con un provvedimento che ha, come motivazione e giustificazione, un errore redazionale. Ripeto, credo si ponga una questione di dignità e di rispetto delle istituzioni, perché non è possibile immaginare che si possa affrontare un dibattito su un tema così delicato con una motivazione così indecorosa e così irrispettosa per la serietà delle istituzioni In secondo luogo, Presidente, ho ascoltato l'intervento del senatore Fuda e, per la verità, ben prima della sua autodifesa l'emendamento, proprio per evitare la personalizzazione, anche perché si sarebbe trattato in ogni caso di un approccio riduttivo rispetto all'importanza del problema e della questione, più che «emendamento più che «emendamento Fuda», «emendamento fuga»: in realtà, si tratta di un tentativo per cercare di concretizzare una fuga dalla responsabilità contabile

Signor Presidente, è veramente paradossale che all'interno di una finanziaria che contiene che si possono definire «griffati», addirittura firmati e sottoscritti *a latere*, non si riesca a venire a capo della responsabilità politica relativa all'introduzione di questo comma. Mi sembra francamente una questione che merita un approfondimento, sul quale non dico altro perché so che il collega Storace ha presentato emendamenti in tal senso, che peraltro vanno anche nella direzione indicata dal collega Saro per determinare chiarezza e trasparenza rispetto a questo dato e a questo elemento. Aggiungo ulteriormente che non vi che non vi è solo il problema di una finanziaria con emendamenti chiaramente attribuibili, anche rispetto agli interessi oltre che alla fonte di scrittura della norma, ma vi è un problema più ampio di carattere politico. Questa vicenda si inserisce in un contesto che, soprattutto sul terreno locale ed amministrativo, disegna un quadro dove stiamo ritornando in una condizione di prevalenza della illegalità e della cultura delle impunità. Questo emendamento non è un incidente di percorso. Si inserisce all'interno di una condizione che vede ritornare un meccanismo per il quale la cultura dell'impunità è tornata ad essere prevalente. Allora buonsenso, capacità di affrontare correttamente le questioni ed i problemi avrebbero suggerito e suggerirebbero la riflessione su questi temi all'interno di un ridisegno organico del sistema a partire dal sistema degli enti locali nel recupero di un diverso equilibrio tra poteri, responsabilità e controlli anche perché in questo meccanismo che si è instaurato nel corso degli anni, il degrado della politica e dello spirito pubblico, quello della Corte dei conti è restato l'unico caposaldo in termini di controlli per evitare evitare che si torni ad un meccanismo per cui siano le aule giudiziarie a risolvere i problemi che la politica ed il dibattito politico non riescono a fare. Quindi, non è possibile affrontare questo tema con con l'ipocrisia emersa di questi falsi moralisti, i quali non hanno il coraggio, quale primo elemento di moralità dell'assunzione della responsabilità politica.

distogliere le responsabilità che il Governo ha avuto in tale questione. Però la verità, colleghi, credo sia evidente: qualcuno ha cercato di fare il furbo; non c'è riuscito, la frittata è stata fatta. Prendiamone atto, anche senza eccessivi drammi. Da parte nostra rinunciamo a strumentalizzare tale questione, che sicuramente la sinistra avrebbe ingigantito nel modo più assoluto a parti invertite. Però, per favore, non tentate di dare la responsabilità di tutto ciò a noi. Se è vero che ci siamo opposti allo stralcio di questa norma, ciò è avvenuto non certo perché eravamo d'accordo con la stessa, ma perché volevamo che il Governo si assumesse fino in fondo la responsabilità politica di quanto accaduto. C'è il furbetto del quartierino anche all'interno del Governo. È del tutto evidente che una norma così dirompente non non essere stata dettata da un Ministro. È assolutamente evidente, colleghi, dobbiamo prenderne atto; e bisognerà pure che ben salti fuori, prima o poi, il nome del furbetto, credo che sia interesse anche e soprattutto del Governo, altrimenti il sospetto

colleghi, il Ministero della giustizia, sotto la mia guida, ha accumulato circa 100 procedimenti per danno erariale (non so se sia un *record* nella storia della Repubblica, probabilmente sì), di cui 75 in capo al sottoscritto. Bene, nessuno di essi riguarda l'emendamento Fuda. I procedimenti cui il sottoscritto e tutti gli altri miei collaboratori al Ministero della giustizia sono sottoposti non vengono salvati da tale emendamento, poi trasformato in articolo. Quindi, non parlo per interesse personale; credo che vada detto per chiarezza. Detto ciò, mi sembra che un bene sia nato da tale vicenda, e lo hanno sottolineato molto oratori intervenuti prima di me: occorre focalizzare come lavora la Corte dei conti. Credo che il Parlamento debba in qualche modo intervenire per sanare quello che oggi è un vero e proprio malfunzionamento che, da un lato, fa crescere e aumentare enormemente il contenzioso pendente e, dall'altro, comporta soprattutto una vera e propria ingiustizia nei confronti degli amministratori. degli amministratori. Vedete, è del tutto logico che un amministratore debba essere sottoposto al controllo di un organo, che tra l'altro ha valenza costituzionale; su questo non ci piove, però bisogna vedere le modalità, e soprattutto un amministratore deve sapere, in maniera assolutamente chiara, quali sono i limiti entro i quali può operare. Per saperlo non c'è allora che un modo: ci devono essere procedimenti rapidi, in modo che vi sia una giurisprudenza che fa scuola, ma soprattutto in modo che l'amministratore possa sapere rapidamente se ha agito male o in maniera corretta. Invece oggi cosa accade? Accade che la Corte dei conti, lo dei conti, lo vediamo ogni anno, bacchetta tutti. C'è la relazione del Presidente, che parla *ex cathedra*, che dà il voto a tutti: agli organi di Governo, alla finanziaria, all'economia.

è? I provvedimenti giacciono anni ed anni. Bene, questo non deve più accadere. È allora del tutto evidente che noi voteremo a favore della soppressione di quell'articolo, perché è una strada sbagliatissima. è cercato con un sotterfugio di risolvere un problema che invece è reale: quello, ripeto, da un lato, della possibilità degli amministratori di operare e, dall'altro, se hanno sbagliato, di poter vedere riconosciuta o

medaglie più negative c'è sempre il lato positivo: l'aspetto positivo è che oggi venga alla luce e venga dibattuto per la prima volta questo problema in Parlamento. Poi, per favore, colleghi, smettiamola noi politici di avere la coda di paglia nei confronti degli altri organi dello Stato.

la mia capacità e la mia onestà, così come quella di tutti. Dobbiamo avere la forza di legiferare su questi temi senza aver paura di attacchi strumentali da parte di nessuno. Se il Parlamento non si da questo stato di sudditanza rispetto ad altri organi e poteri dello Stato non riusciremo mai a legiferare nell'interesse del Paese. Questo è il messaggio forte che dobbiamo lanciare da quest'Aula approfittando di tale problema.

inosservato. Dobbiamo uscire da quest'Aula con l'impegno ad affrontare seriamente questa materia, perché chi amministra e fa politica ha il diritto di sapere in tempi ragionevoli se ha operato per il bene del Paese o se in qualche caso ha sbagliato e, in questo caso, affrontare la giusta condanna. ancora per un minuto per dire una cosa importantissima. Con tutta la modestia possibile, io ritengo che la lettera del procuratore sia sbagliata.

Diamo per scontato che quando si fa una finanziaria così complicata come l'ultima che abbiamo esaminato in Aula al Senato (o che abbiamo finto di esaminare) può anche infilarsi qualche comma in modo imprevedibile, ma dubito che esso si infili senza sapere chi lo ha voluto.

gli amministratori pubblici. Questo è il senso. Riducendo la durata della possibile prescrizione, riduce la possibilità di sottoposizione al giudizio contabile. Se avessimo discusso di questo comma dieci anni fa probabilmente ce ne saremmo occupati molto poco. Dieci o Dieci o quindici anni fa era molto più evidente la giurisdizione penale in materia di responsabilità degli amministratori, pubblici e locali in particolare. La magistratura penale finiva con il rappresentare una sorta di ultima frontiera, dopo che erano venute meno le frontiere della selezione della classe dirigente amministrativa e politica locale da parte dei partiti politici e dopo che era venuta meno la rete di protezione dei controlli di legittimità, che molto tempo fa servivano a qualcosa e poi, progressivamente, sono andati perdendo di significato, fino, addirittura, ad essere aboliti del tutto. Siamo, quindi, in presenza di un comma della finanziaria che colpisce la sola frontiera che ancora, in qualche misura, regge sulla responsabilità degli amministratori pubblici e locali in particolare. Questa è la gravità della questione. Questo è il punto sul quale il collega Viespoli ha voluto richiamare l'attenzione. Questo è il motivo per il quale, sebbene siamo tutti favorevoli ad abrogare questo comma come come orrendo, siamo preoccupati per il fatto che esso esista. Non siamo preoccupati ovviamente di toglierlo, ma che ci fosse. Le diverse frontiere sulla responsabilità amministrativa erano venute meno, una dopo l'altra. Tanti anni fa è venuta meno l'autorizzazione amministrativa da parte del prefetto, del Ministero dell'interno, caduta per mano della Corte costituzionale in nome dell'autonomia degli enti locali. Poi, in qualche misura, è caduta la responsabilità attraverso i partiti politici, compreso quello dal quale provengo; una responsabilità che si era andata attenuando in funzione del consenso elettorale: non si guardava più in faccia a nessuno che amministrasse, purché avesse il consenso. Poi si è andata attenuando la responsabilità penale. Rimaneva quella contabile, che per molti anni non ha fatto paura quasi a nessuno. Questo comma invece ha visto l'insurrezione dei colleghi magistrati della Corte dei conti perché, come loro perché, come loro hanno dimostrato, si trattava di un comma che avrebbe di fatto ridotto drasticamente la possibilità della responsabilità contabile e/o amministrativa, da questo punto di vista, degli amministratori pubblici, i residui amministratori pubblici nazionali e la stragrande maggioranza di amministratori pubblici locali.

prevalentemente a carico di amministratori pubblici dei partiti che governavano il Paese, i partiti del centro‑sinistra e in particolare quello della Democrazia Cristiana. In questa stagione gran parte degli enti locali è amministrata dal centro‑sinistra. allora, per qualche aspetto ha avuto anche le caratteristiche di un colpo di spugna della maggioranza di Governo sui propri amministratori locali. Vorrei che questo fosse il punto centrale sul quale la maggioranza politica desse risposta. *(Applausi del senatore Storace)*.

sia con mandato politico, sia i tecnici, sono del centro‑sinistra. Possiamo ritenere che una maggioranza politica non sapesse nulla di questo comma? Possiamo ritenere che fosse solo il collega Fuda il responsabile, quando abbiamo emendamenti presentati da una larga quantità di colleghi del centro‑sinistra, compreso il collega Formisano (non so se abbia firmato qualche emendamento senza sapere cosa facesse), molti colleghi vicini a questo o a quell'ex sindaco, di questa o quella città, compresa la città di Roma? Intendo dire: non voglio avanzare sospetti, ma chiedo una valutazione politica da parte dei Gruppi politici del centro-sinistra a carico dei propri amministratori pubblici locali. Questo è un fatto particolarmente grave, non perché io esoneri dalla responsabilità gli amministratori centrali, ovviamente il Governo di centro-sinistra determina ancora di più la possibilità dei propri dirigenti attraverso le forme più o meno varie di *spoils system*. Di questo si tratta, e questa è la ragione per la quale noi riteniamo di dare parere favorevole e quindi il Gruppo dell'UDC voterà, in modo compatto, a favore dell'abrogazione. Ma la ragione per la quale siamo stati notevolmente preoccupati anche noi è che i colleghi della Commissione bilancio non hanno potuto neanche esaminare nel merito questo comma perché, come tutti sappiamo, il cosiddetto maxiemendamento è giunto per la fiducia senza che nessuno sapesse nulla in Commissione. Ecco abbiamo di fronte come un tentativo di colpo di mano; ecco perché non possiamo accettare la spiegazione non solo farisaica, ma vergognosa, che il Governo indica quando presenta il decreto-legge per la conversione, parlando di un mero errore redazionale, quasi si fosse trattato di un fatto tecnico dovuto non si sa a chi.

se ciò è vero, come è stato possibile che la finanziaria sia stata firmata, perché a questo punto è stata firmata con un contenuto contrario all'articolo 81 della Costituzione. è stato risolto dalla stampa (ma giammai dal Governo o da altra comunicazione che sia stata fatta negli organismi parlamentari), nel senso cioè che la firma sarebbe avvenuta contemporaneamente: ma come contemporaneamente? È stata firmata prima la finanziaria? Ma allora questa era

L'unico modo per risolvere la sciarada è che i due provvedimenti siano stati firmati contemporaneamente, uno con la mano destra e l'altro con la sinistra, della qual cosa ringraziamo il Capo dello Stato, anche se ci rimane il dubbio di sapere cosa sia stato firmato con la mano sinistra.

posso dire che non è possibile che in Commissione bilancio si esamini un emendamento o una parte di un maxiemendamento quando non sia stato visitato dagli Uffici. Non solo, ma di ciò si trova traccia (come dicevo poc'anzi

resoconto stenografico, ma in quanto si trattava di un parere ed erano già finiti i lavori della Commissione sulla finanziaria è soltanto un resoconto sommario). Dice infatti il resoconto che il senatore Vegas

in particolare la qualifica di imprenditore agricolo e altre, rilevando che su proposte emendative analoghe contenenti modifiche di tipo ordinamentale il Presidente si è pronunziato nel senso dell'inammissibilità». Sugli emendamenti ordinamentali, del tipo giudiziale, abbiamo svolto un lungo dibattito in Commissione, e in primo luogo sull'emendamento che prevede la possibilità della confisca per alcune ipotesi di reato giudicate già in primo grado e - come per le ipotesi di corruzione era stato aggiunto l'abuso di ufficio - con un emendamento del senatore Castelli e mio questa parte è stata espunta. Per quale motivo la Commissione bilancio del Senato ha continuato a giudicare ammissibili questi emendamenti? Perché in caso contrario avrebbe tenuto un comportamento diverso rispetto a quanto era stato fatto nel corso della finanziaria nell'altro ramo del Parlamento.

Non ci sono, a nostra conoscenza, norme che trovino ospitalità all'interno del testo presentato dal Governo che non hanno un fondamento per materia negli emendamenti presentati»; era stata infatti rilevata l'impossibilità di dare un parere favorevole all'introduzione anche di questa parte.

Voglio però rassicurare il senatore Ferrara in merito alla legittimità di emanare un decreto che interviene sulla finanziaria, che non è ancora

in merito agli effetti che produrrà questa norma che entra in vigore. Devo dire con tutta onestà che pensavamo che da parte del relatore Villone o della sinistra ci fosse una specie di «Abbiamo commesso un grave errore, uno scivolone; non era il caso, *ergo*, ovviamo come possibile», anche se secondo il sottoscritto - e poi lo spiegherò

Non credo che capiti tante volte di discutere un testo normativo che reca una premessa che poi nel corso della discussione generale un membro della stessa maggioranza demolisce, come è successo nel caso Le argomentazioni addotte per presentare questa legge di conversione sono che il famoso comma della finanziaria è stato il frutto di un mero errore redazionale.

qualcosa si può omettere qualcosa o dimenticare, ma una volta che si scrive un comma con questa puntualità, è difficile giustificarlo come un errore redazionale. il senatore Fuda abbia scientificamente spiegato a che cosa finalisticamente era indirizzato viceversa l'emendamento. Era chiaro: si voleva modificare il tempo di partenza della prescrizione dei reati amministrativi contabili, sostituendo causa ed effetto, la condotta con il danno poi prodotto. Chiaramente i tempi sono diversi, si sposterebbe molto in avanti nel tempo il momento da cui parte la la prescrizione e indubbiamente tanti, tanti pubblici amministratori se ne sarebbero potuti avvantaggiare. Abbiamo capito anche che il responsabile della presentazione sembra essere il collega Fuda,

una riunione più ristretta fra referenti di partito: ognuno pone sul tavolo le proprie richieste e si dà poi inizio ad un taglia e cuci. Qualcosa si accetta, qualcosa lo si rifiuta, ma è impossibile che in quella sede emerga qualcosa che non ha a che fare con la discussione politica del momento. Ritengo quindi che lo si sia voluto introdurre. Vengo adesso agli aspetti giuridici, perché parliamo di norme.

criminosa, comunque illegittima, e il momento della sanzione, della sentenza, si accavallano più leggi, c'è una successione di leggi? Interviene un altro principio generale, generalmente accettato

ma successivamente, abrogando quella norma fatidica contenuta nella legge finanziaria. Ciò sta a significare che non può entrare in vigore un minuto prima perché non si può abrogare ciò che non c'è, ciò che non è vigente, non è cogente.

nel momento stesso in cui entra in vigore, ha vigenza ed esplica pertanto tutti i suoi effetti: *ergo*, tutti i giudizi, da quel momento in poi, consentiranno a chi è imputato di avvalersi della norma precedente, della norma intervenuta o della norma abrogata,

saranno inutili. Diciamo pure che siamo d'accordo, però non modificheremo assolutamente nulla, non cambieremo assolutamente nulla. È anche difficile

che è anche difficile esasperare a questo punto i toni nel riprendere tale condotta. Il mio Capogruppo ha già spiegato le motivazioni politiche

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, vorrei sapere, di fronte alla disponibilità dell'opposizione a sostenere l'abrogazione della norma contenuta nella legge finanziaria al comma 1343, se si registra altrettanta disponibilità da parte della maggioranza nel sancire a parole e non solamente con il pensiero che il Governo ha fatto una delle figure peggiori che potesse fare nell'approvazione della legge finanziaria. E dico anche - esporrò i motivi successivamente, nell'intervento che sto svolgendo mi dispiace che non sia presente il vice presidente del Consiglio, onorevole Rutelli, perché la sua sarebbe stata una presenza importante per chiarire alcuni dubbi che abbiamo. Desidero partire dalla relazione del senatore Villone. Quest'ultimo è sembrato quasi imputare all'opposizione il pasticcio combinato dal Governo. Il senatore Villone dimentica che questo pasticcio è stato approvato grazie ad un voto di fiducia che ha blindato la legge finanziaria e che si è voluto impedire una quarta lettura del disegno di legge alla Camera. Sarebbero bastati cinque minuti per

Credo che su tale questione la maggioranza dovrebbe offrire qualche spunto di autocritica al dibattito parlamentare, se non altro per dimostrare buona fede nell'adottare una norma che comunque apprezzo perché elimina il pasticcio che lo stesso Governo ha causato. Questa è una norma approvata in una legge finanziaria per il cui varo è stato determinante, ad esempio, il voto dei senatori a vita, senatori a vita, che hanno consentito che passasse anche questa norma insieme all'obbrobrio caratterizzato dal complesso delle norme della legge finanziaria. Anticipo, signor Presidente, che quando oggi si voterà per le dimissioni del presidente Cossiga forse sarò uno dei pochi ad aderire al suo intendimento di lasciare l'Assemblea del Senato, perché vorrei che le leggi le approvassero i rappresentanti eletti dal popolo. Detto questo, quello che contesto è che non si scriva, nella relazione che accompagna l'approvazione di una norma per abrogarne un'altra, che cosa - senatore Fuda - prevedeva la norma in questione. Credo che qui ci sia davvero un grave difetto di responsabilità da parte della maggioranza che governa - si dice per volontà popolare, anche se abbiamo qualche sensazione contrastante - nel non

la prescrizione decorreva dal momento in cui si verificava il danno, quella norma faceva risalire la prescrizione dal momento dell'approvazione dell'atto, anche se nel frattempo non fossero intervenuti altri eventi. Ebbene, ho ascoltato con molta attenzione, e per la verità con tanta fatica, l'intervento del collega Fuda, che è colui che ha elaborato la norma originaria, almeno su questo possiamo essere d'accordo. Una norma più complicata del discorso che lei, senatore, ha fatto qui e mi dispiace che sia presidente della Commissione per la semplificazione della legislazione perché non abbiamo capito assolutamente nulla delle ragioni che lei ha addotto a sua difesa. Una sola cosa ho capito, senatore Fuda. Lei ha detto: non sono stato io. Ed allora ha ragione o no il presidente D'Onofrio a chiedere chi è stato a fare questo pasticcio? Questo abbiamo il diritto di saperlo proprio per far conoscere al Paese che in quest'Aula non ci sono persone che hanno voluto favorire qualcun altro. Credo che sia un atto importante e per questo abbiamo anche presentato alcuni emendamenti specifici tra quelli che si sono salvati dalla tagliola del Presidente delle Senato (che ho accettato, pur contestandola e subendola), perché vogliamo sapere, riguarda gli emendamenti, se ci sarà disponibilità da parte della maggioranza nel dare un segnale alla pubblica opinione di voler fare realmente trasparenza, nel senso di non mettere sotto il tappeto la spazzatura che si trova e dire che è stato Tizio o è stato Caio e che ne avrebbe beneficiato Sempronio. Se non si fa questo, il problema della responsabilità di chi ha ordito questa manovra ve lo porterete appresso ogni volta che parleremo di tali questioni. Vede, Presidente, io mi sarei aspettato, nel momento in cui il Senato riceve il testo da parte del Governo, una segnalazione all'Esecutivo almeno sulla relazione che accompagna la norma. Già ne ha parlato eloquentemente il collega senatore Viespoli e lo ha ribadito anche il senatore Divina: non si può scrivere una bugia su un atto che viene sottoposto all'approvazione del Parlamento. Non è vero che c'è stato un mero errore redazionale, c'è un stato un gravissimo orrore politico, una manovra per favorire qualcuno. Io credo che ci voglia onestà da parte di tutti nell'ammettere questa considerazione nel dibattito. Noi abbiamo alcune preoccupazioni, Presidente, che voglio rassegnare all'Aula: alcune di queste erano contenute negli emendamenti che avevo proposto e che sono stati cassati dalla Presidenza del Senato,

che la firma del decreto, successiva alla firma della finanziaria, non comporti effetti e qualche avvocato non possa avere ragione nel sostenere il principio del *favor rei* nella difesa del proprio assistito. Siamo sicuri che gli stessi tempi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, prima la finanziaria, poi ovviamente il decreto che abroga una norma, non possano aprire una finestra all'interno della quale agitare contenziosi e conflitti che vadano poi a cassare Si tratta di una questione di assoluta importanza sulla quale sarebbe bene fare chiarezza da parte del legislatore. Poi ci sono i problemi più eminentemente politici, non intervengo su quelli di carattere giuridico. avvenute, a seguito dell'approvazione della finanziaria, alcune questioni, e per questo avrei voluto qui la presenza del Vice presidente del Consiglio, sulle quali il Senato ha il diritto di esigere chiarezza. fanno parte di altri due emendamenti cassati che ho trasformato in ordini del giorno, che riguardano segnatamente iniziative annunciate dal Ministro delle infrastrutture e dal Vice presidente del Consiglio con delega ai beni culturali. Il ministro di Pietro, e non oso dubitare che non abbia dato seguito alla propria azione, ha annunciato di aver segnalato alla procura della Repubblica di Roma il caso in questione, chiedendo che si aprisse un fascicolo. Vorrei sapere se questo è stato fatto e se il Governo non intenda sostenere a propria difesa l'azione meritoria del ministro Di Pietro che chiede di fare chiarezza sulle riunioni che hanno determinato la stesura e l'approvazione successiva da parte del Governo della proposta al Consiglio dei ministri. L'altra questione che vorrei si faccia capire al vice Presidente del Consiglio riguarda il fatto che i dubbi sollevati dalla stampa non possono essere demonizzati a colpi di querela.

ma non è assolutamente giustificabile il livore nei confronti de «Il Giornale» che ha posto dubbi sulla condotta o di Rutelli o del suo partito in questa vicenda. Il Vice presidente del Consiglio, anziché querelare «Il Giornale», anziché minacciare ghiotti risarcimenti pecuniari o la galera nei confronti dei giornalisti, avrebbe il dovere di venire in Senato e dirci chi è stato a fare questa manovra, perché altrimenti vuol dire che si può coprire tutto, approviamo il decreto, nessuno deve sapere nulla. Noi vogliamo saperlo perché alla fine, Presidente, sa cosa rischia di succedere? Che l'unico che paga in questa vicenda è un redattore de «Il Giornale» che si è permesso di avanzare dei dubbi, e questo non è giusto in una democrazia. Vogliamo anche che il Vice presidente del Consiglio risponda ad alcune domande. Noi abbiamo presentato un'interrogazione al Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, al vice Presidente del Consiglio, ai Ministri dell'economia, della giustizia e delle infrastrutture alla quale il Governo si è ben guardato dal rispondere. Vorrei sapere se verrà mai il momento in cui il Governo risponderà a domande impegnative. Resto sul tema sollevato dal vice presidente del Consiglio Rutelli nei confronti del quotidiano «il Giornale» sulla questione del comma 1343 della finanziaria: ho chiesto se fosse a conoscenza di questo emendamento presentato da un collega del suo partito; se fosse a conoscenza del fatto che l'emendamento in questione era stato presentato anche alla Camera da un deputato del partito della Margherita; se fosse a conoscenza che l'emendamento è stato presentato qui al Senato l'8 dicembre scorso e non portava solo la firma del senatore Fuda ma anche del Vice presidente del Gruppo dell'Ulivo e da altri autorevoli esponenti della Margherita. Vogliamo sapere se sono stati delegati dal vice presidente Rutelli esponenti del suo partito a condurre la trattativa in sede di stesura del maxiemendamento alla finanziaria;

e, infine, se non intenda sostenere l'azione del ministro Di Pietro nei confronti della procura della Repubblica di Roma. Di fronte a simili domande, si oppone un silenzio che preoccupa la pubblica opinione, la quale ha diritto di sapere chi si sarebbe avvantaggiato da questa norma. Signor Presidente, non sono solamente io a parlare di manina che ha infilato, non per mero errore materiale, ma per precisa volontà politica, il cosiddetto emendamento Fuda all'interno della legge finanziaria;

più importante che abbia tenuto il centro-sinistra da qualche tempo a questa parte, che si sta cercando il mandante? Mi domando inoltre se noi dovremmo approvare a scatola chiusa un decreto senza sapere qual è l'impegno reale del Governo a verificare chi è stato l'uomo, il soggetto, la combriccola che ha dato vita a questo autentico pasticcio.

è una questione importante ed è esattamente la domanda politica che ha posto il presidente D'Onofrio e che faccio mia. Vogliamo sapere nomi e cognomi delle persone che si sarebbero avvantaggiate nel caso fosse entrata in vigore la cosiddetta

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, credo che su questo tema siano necessarie alcune considerazioni più di metodo che di merito. I colleghi ne hanno già parlato, il lungo il lungo intervento introduttivo del collega Fuda ha tentato di spiegare come il comma comma 1343 introdotto nella finanziaria faceva in realtà parte di un contesto più ampio, sul cui merito si può discutere, ma che certamente è stato in qualche modo stravolto

discutere. Il testo della finanziaria che questo decreto-legge vuole modificare è assolutamente inaccettabile;

quanto sposterebbe i termini di prescrizione così indietro da rendere vana qualsiasi azione diretta a perseguire gli illeciti contabili non solo per i procedimenti pendenti, ma chissà per quanti anni per i procedimenti a venire. Diciamo la verità: non abbiamo certo bisogno di una norma di amnistia generalizzata come questa, perché sappiamo, leggiamo, verifichiamo, sentiamo ogni giorno che vi è una degenerazione continua nell'attività di esercizio dei poteri pubblici nell'ambito della pubblica amministrazione a livello locale, regionale e, perché no, anche statale. no, anche statale. Quel che mi preme riprendere nel mio breve intervento è la questione del metodo. Questa mattina, intervenendo in apertura di seduta, ho definito il comma 1343 come il frutto avvelenato della finanziaria, ma soprattutto di un modo di procedere dei lavori parlamentari che è degenerato sempre più, sino a toccare il vertice assoluto con la legge finanziaria licenziata a dicembre. ricordo ai colleghi, il presidente Marini, in occasione della presentazione del maxiemendamento, richiamò la decisione della Giunta sulla valenza del voto di fiducia e quindi affermò che, in base a quella deliberazione, qualsiasi esame preventivo del maxiemendamento fosse precluso, feci presente che quella deliberazione risaliva ad oltre 20 prima, in un sistema politico e parlamentare che non avrebbe minimamente immaginato che si potesse arrivare a questi esiti, nonché ad altri, pur meno gravi, che hanno preceduto la finanziaria del 2007.

da condividere, ma di fronte a situazioni che certamente non potevano avere il peso, l'incidenza e l'invadenza di quella rappresentata in maniera esemplare dall'ultima finanziaria.

ma è soprattutto un problema di verifica dell'applicazione dei Regolamenti che ci sono, se certe formule presenti nel passato non siano più

rappresentato pubblicamente, in maniera ferma, soprattutto per chi conosce a fondo simili problematiche, che il maxiemendamento,

ma non sono solo questi i comportamenti anomali. Ve ne sono tanti altri. Per prevenirli è necessario, non solo un lavoro da parte della Commissione affari costituzionali, o della Commissione affari costituzionali

nel momento in cui si presenta un maxiemendamento al Senato, per il fatto che sullo stesso vi sia la fiducia, qualsiasi tipo di verifica sia preclusa, perché questa è la conseguenza cui ha portato la delibera della Giunta. Ricordiamoci che l'incarico affidato alla Commissione bilancio di una lettura del maxiemendamento è stato dato quasi *extra ordinem*, cioè al di fuori di canoni che si potevano invece rinvenire nella delibera di Giunta. È stata cioè affidata alla Commissione bilancio Chiedo allora, nell'interesse dell'istituzione Parlamento, che su questo problema si proceda ad una discussione chiara, ad un approfondimento sereno e forte per arrivare a stabilire il seguente principio: anche di fronte ad atti sui quali vi è la fiducia da parte del Governo,

assoluta di questa vicenda. Cari colleghi, per arrivare alla vicenda in esame, mi corre l'obbligo di dire due parole su come si è arrivati all'inserimento di questo pezzo nella finanziaria, dovuto soprattutto a procedure che tutti quanti giudichiamo inammissibili ma che, se vogliamo essere creduti, dobbiamo cominciare a valutare per sminare il terreno da certi rischi. Abbiamo apprezzato in Commissione anche il coraggio del sottosegretario Lettieri che ci ha illustrato una letterina sulle vicende del pezzo di finanziaria in questione. Come è stato detto anche da altri colleghi,

alla voce Corte dei conti non è stato messo in evidenza il primo pezzo dell'emendamento che contiene, invece, l'amnistia. Allora, Presidente, è una giustificazione del tutto risibile del tutto risibile sol che si considera che per essere cancellato un pezzo della finanziaria deve esserci qualcuno che ha inserito nel testo il corpo principale dell'emendamento, trasformandolo in un comma della finanziaria. Il problema è chi sia stato questo qualcuno che ha inserito nel corpo del maxiemendamento il testo originario dell'emendamento, oggetto poi di questa riduzione

ancor meno visibile rispetto al comma originario che in qualche maniera ha inserito nel testo della finanziaria. Questo è il punto fondamentale. A me spiace che il Sottosegretario e il Governo, per bocca sua, abbia potuto sostenere una tesi del genere. Vorrei poi aggiungere che il comma unico

una legge che non è la solita leggina che può transitare in queste Aule, della quale magari si perde memoria, che non è rubricata magari pur nelle corpose librerie informatiche di leggi e documenti. No! La legge 14 gennaio 1994, n. 20 è la legge generale sulle competenze della Corte dei conti. Non è una leggina introdotta in una finanziaria di 15 o di 5 anni fa, per cui può essere sfuggita a questo zelante ricercatore di vizi di questo maxiemendamento, formatosi per virtù dello spirito santo! Vorremmo appunto sapere a quale nome e a quale cognome corrisponda questo spirito santo. Quindi, dando atto di tali precedenti devo anche dare atto della correttezza della posizione in Aula delle forze di opposizione. Perché quando ci si danno delle regole - e le regole non sono state date da noi, perché da noi sono state contestate, ma sono state applicate in maniera critica dalla Presidenza - bisogna poi avere il coraggio di affrontare le conseguenze. Una di queste conseguenze era quella di avere il coraggio di approvare il maxiemendamento, di rispedirlo alla Camera, di espungere quel comma e di riportarlo al Senato. Questo è il coraggio delle proprie scelte. Il Senato, Il Senato, la maggioranza e la Presidenza non hanno avuto tale coraggio e oggi ci troviamo con una modifica a una finanziaria fresca di stampa stampa su un argomento estremamente grave e serio, i cui esiti non sappiamo ancora quali potranno essere. Potremmo anche trovarci di fronte a conseguenze estremamente gravi, che si sarebbero potute evitare con una corretta navetta tra Camera e Senato. Questo non è stato voluto e credo che la responsabilità politica e istituzionale sia tutta del centro-sinistra, di questo metodo di governare e di fare le leggi.

di menzogna e di ignoranza e io, a mia volta, l'ho accusato di analfabetismo. Quindi, diciamo, c'è stato uno scambio di piacevolezze che

Non intendevo censurare la Commissione bilancio. Anzi, in un passaggio della mia relazione ho detto che la ristrettezza dei tempi con i quali la Commissione bilancio si è trovata a lavorare non aveva dato modo di approfondire. Quindi, volevo dare atto che lo scontro che c'è stato in realtà nasceva da un equivoco. Poche parole poi nel merito, sul profilo tecnico e sul profilo politico. Abbiamo ampiamente argomentato già in Commissione, e poi qui in Aula i colleghi hanno ripreso gli argomenti esposti, per buona parte.

Nel merito, ho molto apprezzato gli interventi dei colleghi, mi riferisco in particolare agli interventi ampi e argomentati dei colleghi Fuda e Saro, ma confermo la mia lettura, cioè che si trattasse di un'innovazione non accettabile, in quanto tale da modificare profondamente il modello generale della responsabilità. Condivido l'esigenza di dare rapidità

dall'ultimo segmento, quello della prescrizione, è il modo sbagliato per farlo. Non possiamo indebolire e rendere evanescente il quadro della responsabilità di chi amministra. È una questione di sistema, lo dicevano, tra gli altri, i colleghi D'Onofrio e Storace. Non possiamo quindi intervenire in modo privo di organicità e inconsapevole degli effetti sul complesso del sistema delle responsabilità. Infine, sul profilo politico, concludo con questo. Mi è stato detto che ho cercato di occultare le responsabilità dell'inserimento di questo comma. Il collega Viespoli ha fatto anche qualche battuta a questo proposito. Io non credo affatto di aver cercato di occultare alcunché. Ribadisco che rifiuto di colpevolizzare i colleghi che hanno preso l'iniziativa. censuro, come ho detto, che questo emendamento sia entrato nella finanziaria nonostante un'esplicita manifestazione di volontà in senso contrario della maggioranza. Noi non dovremmo essere qui oggi a discutere, e ne ho dato atto. In questo consiste la responsabilità politica: discutendo oggi di questo decreto, noi facciamo valere una responsabilità politica indiscutibile. Se c'è un decreto, è perché Governo e centro sinistra riconoscono che il comma 1343 non doveva essere nella finanziaria.

Con questo decreto, centro-sinistra e Governo accettano la responsabilità politica e se ne fanno carico. Per questo motivo, posso serenamente confermare la richiesta all'Assemblea di votare a favore

per eliminare le difficoltà che spesso si incontrano e che sia il Governo che il Parlamento hanno incontrato nella legge di bilancio.

Mi soffermo sul primo. Una legge perfezionata non soltanto nella sua approvazione bicamerale ma anche nella sua promulgazione e pubblicazione ufficiale ha vita autonoma. L'efficacia appartiene alla legge come fatto distinto dalla sua formazione. È, dal punto di vista delle fonti normative, un'entità autonoma su cui il Parlamento può ritornare prima ancora che questa legge abbia efficacia, cioè nel termine di *vacatio*. Non esiste molta letteratura al riguardo, ma da quel poco che ho trovato in una ricerca svolta ieri sera emerge che non soltanto non esiste nessun problema dal punto di vista normativo per questo intervento, ma che, ove si dovesse attendere necessariamente l'inizio di efficacia, questo produrrebbe due effetti, entrambi nefasti. In primo luogo le conseguenze negative avrebbero un inizio in questo caso estremamente preoccupante e pericoloso. In secondo luogo, il Parlamento sarebbe privato del potere di ritornare sui suoi passi immediatamente, e prima ancora della intervenuta efficacia della legge stessa. I

né forti implicazioni all'interpretazione che la stessa Corte dei conti dovrà dare circa l'operatività del decreto‑legge; un'operatività immediata, con cui il Governo ha dimostrato di essere ben consapevole degli effetti nefasti e pregiudizievoli, comunque estremamente preoccupanti, di questo famoso comma. D'altra parte, anche quanto è stato proposto circa un diverso intervento, che toccasse l'operatività, cioè allungasse nel tempo l'efficacia di questo decreto, per poi intervenire successivamente, ripropone negli stessi termini la possibilità di intervenire su una legge prima ancora della sua efficacia. Tanto vale, allora, adottare un decreto, come ha fatto il Governo, che elimini immediatamente qualunque preoccupazione. Per quanto riguarda l'altro aspetto, più denso di significato politico, non posso che riportarmi a quanto ha riferito in Commissione il sottosegretario Lettieri. Posso aggiungere, sulla base della mia esperienza nel campo e presso l'ufficio legislativo, che è prassi costante che tutti gli emendamenti di maggioranza vengano riportati in un unico *file*, il quale subisce poi la lettura e la purgazione da quello che non deve passare. Quindi è estremamente verosimile quanto indicato nel suo accadimento dal sottosegretario Lettieri. D'altra parte, questo ben può, per i sospetti sollevati dall'opposizione, costituire materia del potere ispettivo che il Parlamento esercita sul Governo, attraverso interrogazioni e interpellanze.

Presidente, gli ordini del giorno sono estremamente sintetici e spero che l'Assemblea e il Governo vogliano apprezzarne le finalità. Mi riferisco prima agli ordini del giorno e per brevità esaurirò

sulle responsabilità esistenti in ordine all'inserimento del comma 1343 nella legge finanziaria 2007. Questa, onorevoli colleghi, è una norma di autotutela del Governo. Da fonti autorevoli dell'Esecutivo, infatti, è venuta l'indicazione - cito il caso del ministro Di Pietro di una manina che ha inserito questo comma. Il ministro Di Pietro ha annunciato la sua segnalazione alla procura della Repubblica di Roma. Proprio perché il Governo si dice irresponsabile di fronte a quanto accaduto o non responsabile e sicuramente non corresponsabile,

vicenda in sé molto complicata, se non altro a risparmiare querele nei confronti dei giornali che hanno riferito su di essa. Credo che, se vi è stato un errore riconosciuto e se vi è stata una manovra che al Governo non era conosciuta, sia legittimo il dubbio che possono aver avuto alcuni quotidiani. Chiediamo al Governo di evitare di trascinare in tribunale giornalisti che hanno sollevato dubbi, anche se fossero i più duri. Si tratta, infatti, di una vicenda che ha costretto il Parlamento a legiferare di nuovo, quindi almeno il dubbio era ammesso. Chiediamo al Governo di farsi carico di una licenza del diritto di cronaca, che non penso possa essere messa in discussione dal comma che oggi ci accingiamo ad abrogare. Infine, per quanto riguarda gli emendamenti, sono due quelli che sono stati ammessi dalla Presidenza; anch'essi si riferiscono alle responsabilità. L'emendamento 1.101 fa riferimento alla necessità che il Governo riferisca al Parlamento,

Presidente? Non tutti i senatori sanno cosa ha detto il sottosegretario Lettieri in Commissione, ma sarebbe auspicabile, sottosegretario Scotti, che il Governo conducesse una propria inchiesta e riferisse sull'esito della stessa al Parlamento, proprio per sgombrare i dubbi sulla buona fede dell'Esecutivo. Il successivo emendamento 1.102 invita il Governo, proprio perché si dice serio di fronte alla questione, a fornire i nomi di chi avrebbe beneficiato della norma, per capire anche se è vero il pandemonio che si è creato dopo l'introduzione del comma Fuda all'interno della finanziaria.

e 2.101, i quali ad una successiva rilettura appaiono tecnicamente sbagliati perché porterebbero ad un risultato esattamente opposto a quello che ci prefiguravamo, cioè manterrebbero in vigore

pena poi la prescrizione. Colleghi, non è così: i cinque anni riguardano esclusivamente il tempo a disposizione della procura per aprire il procedimento di responsabilità di danno erariale, ma una volta che esso è aperto non c'è più prescrizione, la causa può andare avanti eternamente. Ci sono cause che sono durate 25 anni, per 25 anni un amministratore non ha potuto sapere se era colpevole o no, se dovesse risarcire oppure no. Ricordo che addirittura esiste una norma per la quale il danno erariale si trasmette agli eredi, si trasmette agli eredi, per cui eredi assolutamente incolpevoli potrebbero essere chiamati a rispondere di un danno che ha compiuto il proprio padre o comunque colui il quale ha lasciato loro l'eredità. Credo che questo sia veramente un caso di inciviltà giuridica. Questi emendamenti, dunque, si propongono semplicemente di stabilire un termine ragionevole di prescrizione entro il quale la Corte dei conti debba portare a termine la sentenza.

può tecnicamente di certo fare. Quindi, su questo mi rimetto alla valutazione del Governo. Ritengo invece di esprimere parere contrario sull'ordine

La denuncia o la querela può essere presentata dal singolo componente del Governo a titolo individuale, ed il Governo non può né impedire questo né chiedere al singolo componente di fare una denuncia o una querela. Non è pensabile, per intenderci lo dico come esempio - che il Presidente del Consiglio dei ministri faccia una denuncia o una querela previa delibera del Consiglio dei ministri; se fa ciò, interviene a titolo

proposte: togliere le cause della interruzione della prescrizione e allungare il termine di prescrizione al fine di dare certezza. Come ho già detto in precedenza, condivido l'esigenza di dare rapidità al giudizio della Corte dei conti, conti, ma personalmente sono contrario ad interventi che rompano con il modello generale della responsabilità e dell'azione di risarcimento del danno; fatto che questi emendamenti sicuramente creano, in quanto le cause di interruzione della prescrizione sono elemento costitutivo del modello generale dell'azione di responsabilità. Non possiamo - credo - in questa sede, in maniera così parcellizzata, fare un intervento di sicuro rilievo sistematico che

il primo presentato si intende dire che l'Avvocatura dello Stato nella sua autonomia istituzionale e obiettività debba dare debba dare il suo contributo professionale alla procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati (ove ci fossero, ove ci siano e ci saranno), lo si può accogliere senz'altro come raccomandazione.

nel senso cioè che è preferibile lasciare che anche la stampa esprima la propria opinione senza poi doversi sentire la spada di Damocle di una eventuale denuncia. Tuttavia, non è possibile che il Governo si possa impegnare a tanto.

spuri rispetto all'oggetto del decreto-legge e su questi esprimo parere negativo. Altri ancora possono essere trasformati in richieste di esercizio del potere ispettivo del Parlamento attraverso interrogazioni attraverso interrogazioni e interpellanze. Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Castelli, il fatto che si allunghi la prescrizione per uno o dieci anni oppure la si interrompa in determinati casi può provocare una duplice conseguenza: per un verso, un contrasto con l'articolo 111 della Costituzione proprio in un tempo in cui il Dicastero della giustizia, comunque l'intero Governo, si propone di ridurre i tempi della giustizia e, quindi, anche di quella contabile; per altro verso, una difformità

*relatore*. Comprendo benissimo il senso degli argomenti del collega Storace, ma il punto è il seguente: il nostro interlocutore è il Governo, quindi correttamente la Presidenza dell'Assemblea ha fatto scrivere «il Governo».

può impedire né pretendere che i suoi membri facciano o non facciano alcunché nell'esercizio del potere di denuncia e di querela, perché questa è una facoltà

Egli ha posto all'attenzione dell'Aula una questione sulla quale è del tutto evidente la necessità di intervenire e legiferare. Soprattutto ha detto all'Aula - mi sono appuntato i termini che ha usato il presidente Fuda, nei confronti del quale nutro il massimo rispetto

è arrivato persino a dire: «il comma Fuda non mi appartiene» e dal testo del suo intervento, dal contesto e da tutto ciò che ci ha spiegato si capisce che intendeva, intende e intenderà porre all'attenzione delle forze politiche e del legislatore una questione che ha validità scientifica e culturale. Ma, proprio per quel che è avvenuto, è necessario che il Senato faccia un passo avanti. Abbiamo il dovere di tutelare un senatore che dice: «quelle modalità, non mi appartengono, io sono estraneo a quelle modalità, il comma Fuda non mi appartiene». Ebbene, in alcuni degli emendamenti presentati dal senatore Storace c'è un sincero tentativo di scoprire cosa sia avvenuto al di fuori di quest'Aula. Lo dico con chiarezza. Rispetto a tale tentativo noi dell'Italia dei Valori riteniamo che l'Aula

Dobbiamo essere certi di sapere, dopo aver individuato quale è stata la procedura attraverso la quale è potuto capitare che un senatore che è stato sui giornali per dieci giorni abbia potuto dire in quest'Aula «il comma Fuda non mi appartiene e le modalità mi sono estranee», che per il futuro ciò

sulle origini di tale norma. Il senatore Fuda, al quale ho fatto anche le mie congratulazioni questa mattina per il suo intervento, ha sempre detto e chiarito - e per quanto ho potuto seguire personalmente la vicenda le cose sono andate esattamente nei termini che egli ha indicato di aver presentato un altro testo e di non avere più avuto alcun ruolo nella fase successiva. Oggi il Governo è stato silente su questo tema, ancorché interpellato dai parlamentari dell'opposizione.

«Intervenuta la determinazione di espungere dal testo già elaborato le norme sulla prescrizione della responsabilità amministrativa, si è proceduto ad una ricerca informatica». Quindi, è intervenuta ad un certo momento la determinazione di espungere dal testo già elaborato dal Governo quella normativa. Quindi, il testo elaborato dal Governo conteneva quella norma. Successivamente, è intervenuta la determinazione di espungerla e pare che non sia stato possibile. Credo che il Parlamento abbia il sacrosanto diritto di sapere di più su questa vicenda. Piuttosto che attraverso le vie giudiziarie forse il ministro Di Pietro avrebbe fatto bene a porre la questione all'interno dell'Esecutivo di cui fa parte, ma credo che sia doveroso che il Senato, in una vicenda che lo ha visto